Signor Presidente, il Ministero dell'ambiente è impegnato da anni sul tema delle micro e macroplastiche disperse in mare, in anticipo anche rispetto al livello che la discussione ha assunto negli ultimi tempi. È un impegno che si inquadra entro gli accordi internazionali, in particolare quelli sulla conservazione dei cetacei in area Pelagos, l'area pilota dell'accordo Accobams e degli ecosistemi marini, in attuazione degli adempimenti di altri accordi internazionali e nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia marina. Già nel 2007, infatti, il Ministero ha ottenuto l'inserimento della tematica dell'impatto tossicologico delle micro e delle macroplastiche sui mammiferi marini nel Work programme 2008-2010 dello stesso accordo Accobams. Nel 2011 furono stanziati i fondi per i primi progetti scientifici, aventi quale soggetto capofila l'Università di Siena (altamente qualificata e riconosciuta), di monitoraggio e «ricerca orientata», volti alla conoscenza e alla valutazione scientifica di individuazione di metodiche *standard* del fenomeno su scala nazionale e internazionale. I risultati acquisiti nel corso di queste iniziative, ormai indietro nel tempo, hanno consentito più recentemente di sovrapporre la mappa dell'abbondanza delle microplastiche nel Santuario Pelagos, con l'osservazione ed il campionamento dei cetacei, alle mappe della circolazione oceanica. Ciò ha permesso di identificare le cosiddette aree *hot-spot* di accumulo di microplastiche che si sovrappongono in parte alle aree di foraggiamento e di osservazione di esemplari di balenottera comune e delle altre specie di mammiferi marini tursiope e stenella - ed hanno altresì permesso per la prima volta, su scala nazionale ed internazionale, di raggiungere una serie di obiettivi e di linee di azione, che sono elencate nella

Pertanto l'esistenza di gyres nell'area del Santuario Pelagos, in particolare nel tratto di mare compreso tra l'Elba, la Corsica e l'isola di Capraia, non soltanto è un evento noto da tempo al Ministero dell'ambiente, ma sono altresì ben note le caratteristiche di dettaglio in termini di composizione e di densità della tipologia di *marine litter* in esso presente, così come la sua estrema variabilità in termini spaziali e temporali connessi agli aspetti meteoclimatici nonché le loro ricadute su specie "sentinella" quali i mammiferi marini. Per quanto riguarda l'impegno del Governo, che è la sostanza dell'interrogazione, in relazione alla pulizia del mare e delle spiagge si rappresenta come siano state poste in atto iniziative importanti nel campo della prevenzione, nel quale il nostro Paese si è tra l'altro sempre posto all'avanguardia, adottando provvedimenti che mettono al bando i sacchetti monouso non compostabili, *cotton fioc*, materiale plastico e le microplastiche nei cosmetici. Il Governo ha inoltre svolto un ruolo attivo e propositivo nell'attuazione del Marine litter action plan della Convenzione di Barcellona in considerazione della natura transfrontaliera del fenomeno, finanziando anche specifici progetti sulla prevenzione delle emissioni del *marine litter* in mare a Paesi mediterranei, quali la Bosnia e il Montenegro, nell'ambito dell'accordo bilaterale tra il Ministero dell'ambiente e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP-MAP). Per quanto riguarda le azioni di rimozione dei rifiuti dalle spiagge e dai fondali marini,

trasmesso per il prosieguo dell'esame al Senato e che ci auguriamo possa contribuire in maniera significativa, con ulteriori contributi che verranno dalla discussione al Senato, alla riduzione dei rifiuti presenti sui fondali marini in quanto si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati, incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e promuovere l'economia circolare, mediante disposizioni volte a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti accidentalmente pescati o raccolti nella campagna di pulizia del mare e incentivare la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla materia. Nei programmi di monitoraggio all'interno della direttiva quadro della strategia marina che il Ministero dell'ambiente dal 2015 conduce e finanzia, c'è un grande impegno che è stato posto per la valutazione delle quantità dei rifiuti di vario genere presenti in mare. Sono state pertanto svolte indagini accurate e diffuse sui rifiuti spiaggiati, indagando 58 aree distribuite lungo le coste italiane e poste in corrispondenza di foci fluviali, porti, città e aree protette (alla risposta è allegata anche una piantina di dettaglio), sui microrifiuti galleggianti, prelevando campioni lungo transetti fissati da 0,5 a 6 miglia dalla costa in 51 zone differenti, e sui rifiuti presenti sui fondali marini. Questa azione è stata promossa dal Ministero Le indagini sono state svolte principalmente dalle 15 ARPA costiere e organizzate dalle tre sottoregioni marine italiane previste dalla direttiva sulla strategia marina (Mediterraneo occidentale, Ionio, Mediterraneo centrale e Adriatico), utilizzando sempre modalità operative comuni e condivise attraverso specifiche attività di formazione degli operatori. I risultati di queste indagini confermano, dati alla mano, che i rifiuti presenti sulle spiagge sono rappresentati soprattutto da plastica e sono principalmente riconducibili alle categorie cannucce, posate, piatti, bicchieri e sacchetti di *snack* e che le concentrazioni di microrifiuti in mare sono rilevanti tanto sottocosta che al largo in tutti i mari italiani. Per affrontare in modo decisivo il problema, in aggiunta alle misure già dette, alle normative esistenti e a quelle *in itinere*, sono state messe a punto tre misure che consistono nell'individuazione e attuazione di azioni mirate mirate a migliorare la gestione dei rifiuti in relazione all'attività di pesca e acquacoltura, compreso il riciclaggio delle reti, l'identificazione e la creazione di una catena di raccolta e di smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati dai pescatori e anche azioni di sensibilizzazione pubblica (mi riferisco anche alle cose già dette sul cosiddetto In particolare, però, il Ministero sta predisponendo degli accordi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul fondale in alcuni porti selezionati. Questi accordi coinvolgeranno le aree marine protette, le autorità portuali, i Comuni, le associazioni ambientaliste, le associazioni della pesca e quelle della subacquea. Sempre dell'ambito dell'Unione europea, infine, il Ministero opera attivamente affinché le revisioni in corso della direttiva sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico consentano un'adeguata soluzione all'esigenza di mobilitare il mondo della pesca nell'attività e smaltimento della raccolta in mare dei rifiuti e delle modalità di loro corretto smaltimento.

a partire dal tema del disegno di legge salvamare. Nel frattempo, è intervenuta anche la direttiva europea che porterà all'eliminazione della plastica monouso, quindi credo che

alcuni interventi specifici su aree selezionate, con il coinvolgimento delle autorità portuali, delle autorità locali e delle associazioni che si occupano della tutela dell'ambiente e del mare in modo specifico. Credo che il percorso che abbiamo di fronte non sia né semplice, né breve, ma credo anche che il nostro Paese abbia imboccato una direzione corretta che penso possa essere di esempio per altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Signor Presidente, senatrici e senatori, con il presente atto parlamentare l'onorevole senatore interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla categoria dei lavoratori assistenti bagnanti che lavorano alle dipendenze di imprese, cooperative o consorzi che forniscono il servizio di salvataggio ad uno stabilimento balneare, per i quali, a parere dell'interrogante, non è stata riconosciuta la possibilità di accedere alle misure di sostegno messe in campo dal Governo per sopperire all'emergenza Covid-19. Al riguardo devo innanzitutto sottolineare che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fin dall'inizio della pandemia, ha agito per assicurare la fruizione e gli strumenti di sostegno al reddito in favore di tutte le categorie dei lavoratori, al fine di contenere gli effetti catastrofici, che la grave pandemia ha generato nel mondo del lavoro. Per tali ragioni, con il decreto-legge n. 18 del 2020 è stato introdotto un articolato sistema di tutele, che comprende, tra l'altro, l'erogazione di indennità in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti operanti in specifici settori produttivi; in particolare, l'articolo 29 prevede misure di sostegno in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. altresì che, con riferimento ai lavoratori stagionali, nella circolare n. 49 del 2020 dell'INPS sono stati individuati i codici Ateco che identificano le attività, che circoscrivono l'ambito di applicazione della tutela dell'articolo 29. però altrettanto vero che il Ministero che rappresento si è tempestivamente attivato, per predisporre un analogo meccanismo di protezione anche in favore di lavoratori stagionali non operanti nei settori e nelle attività riconducibili a quei codici, come ad esempio il settore del turismo e, per tale ragione, non ricompresi tra i destinatari dell'indennità regolata dall'articolo 29, ma rientranti, viceversa, nelle tutele previste dal Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44 del decreto-legge Più precisamente, con il decreto interministeriale del 30 aprile 2020, il Ministero che rappresento ha stanziato 220 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza. L'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto citato ha esteso la platea dei beneficiari del trattamento indennitario ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Il beneficio concesso, pari a 600 euro, dal decreto interministeriale citato e previsto per il mese di marzo, è stato riconosciuto anche per i mesi di aprile e maggio 2020 e per il medesimo importo, ad opera dell'articolo 84, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Segnalo altresì in questa sede che è in fase di predisposizione un decreto interministeriale, che prevede misure in favore dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, che siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad almeno trenta giornate lavorative, e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, non sembrano residuare vuoti di tutela riguardanti gli assistenti bagnanti, che lavorano nel settore del turismo alle dipendenze di società cooperative, espressamente menzionate dall'interrogante.

per la risposta e per avermi rappresentato il quadro ampio e articolato degli interventi del Governo sulle molteplici categorie interessate e toccate da questa crisi. Ho visto che ha riservato alle ultime due righe finali la risposta all'interrogazione e quindi fatico a dirmi soddisfatto, nella misura in cui non mi sembra che sia stata data una risposta sufficientemente convincente.

Quelli che invece svolgono le stesse mansioni, lo stesso lavoro, e che operano nell'ambito del medesimo contratto nazionale, ma non sono assunti dagli stabilimenti balneari, bensì da cooperative, consorzi o aziende terze, non sono stati compresi nell'erogazione di questo sussidio, perché i codici Ateco sono diversi ed evidentemente non è stata guardata la sostanza della professione ma la forma burocratica riassunta nel codice Ateco. Mi pare che ci sia un problema e che di questo problema il Governo farebbe bene Il trattamento iniquo che qualcuno sconta a fronte dello stesso mestiere e delle stesse mansioni che esercitano altri, che invece hanno riconosciuti i loro diritti, dovrebbe essere sanato da un Governo, perché è una questione di giustizia sociale e casi di così evidente ingiustizia ritengo che

Il senatore Taricco ha richiesto notizie in merito allo stato dei lavori di messa in sicurezza del parco del castello di Racconigi. Come correttamente rammentato dal senatore interrogante, il parco è stato chiuso dal direttore del castello stesso, nell'ambito delle proprie prerogative in virtù dell'incarico rivestito, nell'agosto del 2018, a seguito della caduta di un albero ad alto fusto che ha anche causato il parziale crollo del muro di cinta del complesso e l'interruzione della strada comunale contermine a detto muro, interessata dallo schianto, che solo per fortunata casualità non ha comportato danni a persone. La decisione del direttore è stata adottata anche all'esito di un'indagine fitostatica condotta sulle altre alberature del parco, dalla quale è emersa la necessità di far eseguire improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria su alberature ritenute dal tecnico incaricato a rischio di caduta e quindi pericolose per l'incolumità dei lavoratori e dei visitatori del sito museale. Sono inoltre stati eseguiti interventi in somma urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica. Nel momento in cui il direttore del castello di Racconigi ha ritenuto fossero state assicurate la sicurezza e l'agibilità del parco, è stato riaperto al pubblico il 1° giugno del 2019 il cosiddetto primo anello, ovvero la parte del parco più prossima al castello, avente una superficie di circa 80 ettari. I lavori di manutenzione straordinaria sono tuttora in corso, mentre a breve il sito dovrebbe essere restituito alla pubblica fruibilità nella sua interezza, al termine dei lavori. Vorrei sottolineare che l'attività contrattuale pubblica obbliga al rispetto di normative, regolamenti e procedure ed il Polo museale del Piemonte ha dettagliatamente riferito in merito ai lavori effettuati ed alle procedure per il loro affidamento per un importo di circa 50.000 euro. In particolare, sono state previste operazioni su 60 alberature, calibrate a seconda della necessità: abbattimento di alberi a rischio caduta, potature, messa in opera di di tirantature e lavori di pulizia dei percorsi, nonché ulteriori indagini fitostatiche volte ad approfondire la situazione della stabilità e sicurezza degli alberi del parco. Si è ben a conoscenza delle manifestazioni pubbliche rammentate dal senatore interrogante, tra cui un *flash mob* per la riapertura del parco del castello, promosse o comunque fortemente appoggiate dal Comune di Racconigi e dalla Regione Piemonte. Non mi soffermo tuttavia sulla questione, perché un comunicato stampa è stato già pubblicato a tal proposito dal Polo museale del Piemonte in data 17 maggio 2019. In esso, nel dar conto dei lavori effettuati e di quelli ancora da effettuare nel parco del castello, il competente ufficio piemontese ne annunciava la riapertura prossima, cosa poi, come dianzi accennato, puntualmente avvenuta il successivo 1° giugno. Concludo precisando che la manutenzione ordinaria del parco non è mai venuta meno e che il direttore del castello è già stato sollecitato a vigilare sulla corretta esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la riapertura completa del sito, va osservato che a causa della gravissima carenza di personale tecnico che purtroppo caratterizza il Polo museale presso il quale sono presenti solamente due dei 12 funzionari tecnici previsti in organico, il parco di Racconigi condivide gli enormi problemi nella manutenzione di tutti i siti museali afferenti al polo piemontese. In ogni caso, questo Ministero, proprio per dare una soluzione alla diffusa e grave carenza di personale, ha avviato un importante piano di assunzioni che interesserà il triennio 2019-2021 e che si prevede potrà ovviare alle difficoltà degli uffici che operano sul territorio. Questo consentirà il corretto funzionamento dell'ufficio tecnico e si potrà in tal modo completare una parte consistente delle opere necessarie per la conservazione e la messa in sicurezza del parco monumentale, restituendolo al pubblico nella sua magnificenza. Quanto ai rapporti con gli altri enti competenti, in particolare il Comune e la Regione, l'interlocuzione è stata sempre attiva

Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per la rappresentazione dello stato dell'arte. Noi avevamo fatto questa interrogazione nella primavera dell'anno scorso, dopo che, a seguito del crollo che c'era stato nell'autunno del 2018, erano circolate voci che si sarebbe messo a posto il parco e sarebbe stata fatta manutenzione. Nella primavera passata era poi circolata la voce che sarebbe stato messo a disposizione del pubblico soltanto il primo anello e il grosso del parco sarebbe rimasto escluso. Quindi c'era grande preoccupazione sulla prospettiva dell'utilizzo del parco, partendo dalla considerazione che si tratta di uno dei più bei parchi delle regge sabaude, che ha sempre mobilitato grandissimi numeri di visitatori e svolto un ruolo culturale molto importante, e che la ridotta disponibilità di superficie visitabile stava compromettendo l'immagine complessiva di tutto il castello di Racconigi. Ringrazio il Governo e il Ministero per il lavoro che hanno fatto, che va nella direzione giusta. Apprezzo il fatto, come ci è stato comunicato, che a breve sarà aperto alla visita

della ricchezza del parco non sia interrotta perché, se è accaduto ciò che è accaduto nel 2018, è perché probabilmente il livello di manutenzione non era stato adeguato alle necessità del parco. La seconda questione è la

l'interesse del territorio non guarda a chi gestisce il parco e la reggia nel merito, ma ad avere la disponibilità di un bene che ha una straordinaria valenza sia culturale per il territorio che di *appeal* turistico. Ripeto, l'interesse è di averne la disponibilità e la fruibilità piena, perché non è pensabile - come è successo purtroppo in questi due anni e come noi evidenziavamo nella primavera scorsa - che un bene di questa natura sia tolto alla disponibilità del territorio e dei cittadini. Ringrazio il Governo e verificheremo nei prossimi mesi che quanto è stato qui annunciato trovi soluzione positiva.

a oltre un anno dall'offensiva lanciata dal generale Haftar sulla capitale e nonostante la Conferenza di Berlino, la situazione in Libia rimane particolarmente preoccupante. I nuovi equilibri determinatisi sul terreno pongono, ancora una volta, il rischio di una pericolosa *escalation* che avrebbe nuovamente come vittima principale il popolo libico, che già versa in condizioni umanitarie devastanti. La situazione sul terreno continua ad essere resa ancora più complessa dall'ingerenza di attori esterni, che attraverso il costante afflusso di uomini e materiale, in violazione dell'embargo ONU, continuano ad irrigidire le posizioni delle parti contrapposte. L'Italia è sempre stata in prima linea nel sostegno internazionale alla ricerca di una soluzione politica alla crisi libica ed è tra quei Paesi più direttamente esposti agli effetti destabilizzanti, in termini di minaccia terroristica, sicurezza energetica e pressione migratoria. L'impegno dell'Italia per la pace - grazie a lei, Ministro - si è concretizzato in un intenso attivismo diplomatico nei confronti dei diversi attori libici, dei principali *partner* internazionali e regionali e in seno all'Unione europea, come testimoniato dai recenti contatti del Presidente del Consiglio e della Farnesina con il presidente libico Sarraj e con il generale Haftar e, da ultimo, dalla sua recente missione in Turchia lo scorso 19 giugno. Come accennato, l'impegno italiano si è concretizzato anche in ambito europeo, dove il nostro Paese si è assicurato il comando dell'operazione Irini, finalizzata al monitoraggio del rispetto dell'embargo ONU sulle armi. Ministro Luigi Di Maio, alla luce della sua visita di ieri in Libia, le domando se ci sono delle novità interessanti e quali sono le azioni che l'Italia ha intrapreso o intende intraprendere nel prossimo futuro per sostenere gli sforzi dell'ONU per il raggiungimento di un cessate il fuoco, anche in virtù della recente riattivazione del dialogo in seno al comitato militare misto 5+5 e per rilanciare un negoziato

la missione in Libia di ieri aveva l'obiettivo di dare nuovo impulso a un processo che, anche nel pieno dell'epidemia, non si era mai interrotto, ma deve tener conto di sviluppi importanti. La controffensiva delle forze di Tripoli ha spostato la linea del fronte verso Est, lungo la direttrice tra Giufra e Sirte. La missione di ieri è avvenuta in un quadro di massima condivisione con i *partner* europei: ricordo i recenti incontri con i colleghi francese e tedesco. La Libia rimane, soprattutto per noi, una priorità. L'Italia intende tutelare i propri interessi geostrategici, che coincidono con quelli del popolo libico, stremato da anni di scontri. Al presidente Sarraj, al ministro dell'interno Bashagha e al ministro degli esteri Siala ho espresso la preoccupazione che la contesa per il controllo di Sirte, considerata irrinunciabile da entrambe le parti, conduca a un'*escalation* militare, con l'intervento diretto di attori esterni, o che, invece di una tregua, si giunga a un congelamento del conflitto e a una divisione di fatto del Paese. Abbiamo convenuto sulla necessità di un'immediata e completa ripresa della produzione petrolifera, nell'interesse di tutto il popolo libico. Nel confermare il pieno sostegno italiano alle autorità legittime della Libia, ho trasmesso un invito alla moderazione e ho ribadito che l'afflusso di armi in violazione dell'embargo ONU deve cessare. Un ruolo fondamentale può svolgerlo la missione Irini in questo senso; l'Italia è determinata ad assicurare che sia bilanciata e operi con efficacia e imparzialità, in modo da monitorare, rilevare e comunicare tempestivamente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tutte le violazioni. Ho confermato la nostra disponibilità ad assistere il Governo di Tripoli nello sminamento delle aree intorno alla capitale: sono già state troppe le vittime civili. Ho ripetuto che l'unico percorso credibile verso la pace è un accordo inclusivo di tutti gli attori, con la mediazione delle Nazioni Unite. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione la ripresa dei negoziati del comitato militare congiunto 5+5 e ci aspettiamo l'impegno di tutti per un cessate il fuoco. La mia visita in Libia ha permesso anche di fare un tagliando alla cooperazione bilaterale, in particolare in ambito migratorio ed economico. Il presidente Sarraj mi ha consegnato le controproposte di emendamento alla bozza del *memorandum* del 2017. È un risultato importante, cui tenevamo molto. Le nostre richieste di modifica, formulate a seguito di una concertazione tra Ministeri, erano state sottoposte ai libici il 9 febbraio. Ad una prima lettura sembra che il riscontro fornito vada nella giusta direzione, recependo la volontà italiana di rafforzare la tutela dei diritti umani. Confido che il comitato misto possa riunirsi già il 2 luglio per negoziare il testo. Sul versante della cooperazione economica, l'attenzione si è concentrata sui principali progetti che vedono coinvolte aziende italiane. Ho riferito della mia precedente missione ad Ankara e Sarraj ha riconosciuto l'importanza del ruolo turco per la Libia, ma ha sottolineato con convinzione che l'Italia resta un *partner* insostituibile. In questo senso il ruolo svolto dall'Europa è e continua ad essere determinante. Concludo, Presidente: la Libia è per noi sì una questione di sicurezza nazionale, ma riguarda la sicurezza di tutta l'Unione europea. A tal proposito ci faremo promotori di un piano europeo per la ricostruzione della Libia e il rafforzamento delle sue istituzioni, perché riteniamo essenziale che proprio dall'Europa arrivi un segnale chiaro e incisivo nei confronti del popolo libico.

Lei dal suo viaggio in Libia ha portato a casa un risultato importante e non scontato circa il rispetto dei diritti umani dei rifugiati. Infatti, dopo anni di situazioni intollerabili e di assenza di risposte da parte libica, grazie al suo lavoro e alla riconquistata centralità del nostro Paese in Libia, le autorità locali hanno risposto positivamente alla richiesta italiana di modificare il *memorandum* sui migranti. Vorrei ricordare che tale dramma ha origine dalla guerra civile scatenata dal folle intervento armato nel 2011, avallato dal Governo di Forza Italia, Lega e Meloni. *(Applausi)*. Una guerra basata su *fake news* che ha devastato un Paese sovrano, con il quale Berlusconi poco prima aveva stipulato addirittura un trattato di amicizia. Mi auguro che questi gravi errori dei governi passati, che ereditiamo anche in politica estera, possano servire da monito per le crisi future, ricordando sempre che la guerra genera solo destabilizzazioni e quei flussi migratori incontrollati su cui troppo si è speculato nel nostro Paese. Concludo dicendo che, anche se più lunga e tortuosa, la strada del dialogo e della pace, come più volte ci ha ricordato Papa Francesco, è l'unica capace di perseguire risultati duraturi.

Sono convinta che l'effetto recessivo del *lockdown* sull'economia ci dia l'impulso necessario per affrontare una delle riforme più attese e più utili. La riforma fiscale certamente merita di essere posta tra le priorità del Governo e anche nel Piano nazionale delle riforme e questo lei l'ha recentemente confermato, questa riforma, per essere chiamata tale, necessita di essere affrontata nel suo complesso, come ci ha ricordato anche il Governatore della Banca d'Italia recentemente, e non imposta per imposta come il dibattito politico di oggi sembra dimostrare. Il momento economico è davvero molto difficile e noi dobbiamo utilizzare tutte le leve fiscali in nostro possesso. Non siamo all'anno zero, certo, molti provvedimenti sono stati fatti a partire dal cuneo fiscale, a partire dalla cancellazione delle clausole di salvaguardia IVA alla sospensione dei versamenti che hanno dato certamente sollievo alle famiglie e garantito la sopravvivenza di molte imprese, ma nessuno di questi provvedimenti ha innescato una riforma e oggi dobbiamo fare molto di più. Per rilanciare l'Italia una riforma fiscale complessiva è una misura efficacissima, perché ci dà degli strumenti per fissare degli obiettivi strategici, per plasmare i comportamenti sociali e anche per innescare dei mutamenti nell'economia strutturale veramente profondi. Per essere complessiva, una riforma fiscale deve però contemplare un ventaglio di interventi, partire dalle azioni per colpire il sommerso, dalla trasparenza digitale per premiare i contribuenti onesti, dalla messa a terra del *family act* per dare finalmente una fiscalità alle imprese e alle famiglie, dal pensare a misure

che sono coloro che, più di altri, oggi esprimono questa attitudine all'innovazione e alle scelte sostenibili. La domanda generale che, quindi, le voglio porre - nel quesito ha delle domande specifiche da questo punto di vista riguarda quando iniziamo ad affrontare una complessiva riforma fiscale e quali priorità ci diamo. Nella mia mente sono chiare: dobbiamo lavorare sul sommerso; dobbiamo incentivare la trasparenza fiscale dei contribuenti emersi; dobbiamo lavorare subito sulla *tax expenditure* per ridurre la pressione fiscale; dobbiamo dare una risposta a tutte le partite IVA, agli autonomi e dobbiamo fare un ragionamento di equità sulle imprese. Le fondamenta di tutto questo sono un rapporto di reciproca e rinnovata fiducia tra fisco e contribuenti. (*Applausi*).

il quesito che consente di affrontare la questione cruciale che il Governo ha messo al centro del suo programma e che ha iniziato ad avviare anche con provvedimenti concreti. Ricordo che il 1° luglio 16 milioni di lavoratori pagheranno meno tasse sui loro stipendi per effetto del cuneo fiscale e che il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge *family act*, che prevede un meccanismo di riforma importante di una componente decisiva del sistema fiscale per sostenere le famiglie e la genitorialità. Naturalmente, come è evidente a tutti, la crisi del Covid ha interrotto il lavoro in corso sulla riforma fiscale più complessiva, anche se sono stati introdotti nei decreti approvati delle misure importanti in questa direzione e, prima fra tutte, come lei ha ricordato, la scelta di eliminare permanentemente tutte le clausole di salvaguardia che gravavano sui bilanci degli anni successivi. Adesso si tratta di riprendere questo lavoro nel quadro del progetto più generale di rilancio dell'economia che il Governo sta predisponendo e sul quale si è anche confrontato in occasione degli Stati generali.

una riforma fiscale complessiva, che - come lei ha ricordato - si deve giovare anche di un quadro generale di maggiore trasparenza e più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, sul quale l'amministrazione finanziaria è al lavoro con innovazioni importanti basate su procedure telematiche innovative. C'è, quindi, il tema dell'efficientamento della riscossione. proposito, vorrei dire che occorre anche mettere mano al sistema dell'inesigibilità dei crediti, al fine di eliminare dal magazzino dell'agenzia della riscossione partite creditorie per diversi miliardi di euro che sono soltanto nominali e non hanno alcuna concreta e neppur minima possibilità di recupero per liberare risorse per l'attività di riscossione volontaria e coattiva e così concorrere a una progressiva riduzione

di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, che sono i principi di fondo a cui si deve ispirare la riforma fiscale che il Governo italiano intende varare nel quadro di una strategia più ampia di riforme volte a rilanciare la crescita, la produttività la coesione sociale e territoriale del Paese. ampia risposta, che ci indica la strada da percorrere; noi siamo pronti a percorrerla con lei. È un lavoro straordinario, ma sono convinta che sia la nostra grande occasione per ridisegnare il futuro dell'Italia. Le leve fiscali possono fare moltissimo per ridisegnare il nostro futuro. il nostro futuro. Noi il sommerso lo contrastiamo con l'*intelligence* fiscale e lo contrastiamo non confondendolo con l'emerso. I contribuenti emersi sono noti al fisco; possono essere trattati con merito

È una riforma epocale - lo so che le stiamo proponendo una riforma epocale - che si basa davvero su un nuovo e rinnovato rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco. *(Applausi)*.

dal voto favorevole, talvolta determinante, delle opposizioni e quindi anche di Fratelli d'Italia. A fronte di questo atteggiamento di responsabilità, le ricordiamo ancora una volta la chiusura totale da parte del Consiglio; c'è stato un dialogo finto con le opposizioni e nessuna disponibilità ad accogliere i nostri emendamenti, anche quelli ispirati a sicuro buon senso.

Il Presidente del Consiglio si è fatto notare soprattutto per le dirette televisive e per le conferenze stampa a reti unificate in cui brillava per far dimenticare gli errori che aveva appena compiuto il suo Governo. Ricordo che soltanto ieri il presidente Conte ha dovuto prendere atto - perché la realtà è testarda che la cassa integrazione è fallita, nonostante il presidente dell'INPS rimanga al suo posto. Moltissimi italiani ancora non l'hanno vista e moltissimi italiani l'hanno ricevuta con un ritardo intollerabile. L'ultimo sfregio fatto al Senato e al Parlamento è stata la decisione, da parte del Governo, di non comunicare, ma di fare una semplice informativa al Parlamento rispetto alla riunione dell'Eurogruppo; si è rivelata una prova di debolezza da parte del Governo, perché il Presidente, intimorito dal fatto che la sua maggioranza potesse mancare alla chiamata di unità, ha preferito bypassare il confronto con le opposizioni. Questo è un segno di debolezza; lo sappiamo noi, signor Ministro, ma purtroppo lo sanno anche le cancellerie europee e gli investitori internazionali che devono comprare il nostro debito. Pertanto, la domanda è: perché un'ora soltanto di disponibilità da parte del Governo a relazionarsi con il Parlamento e nove o dieci giorni di Stati generali? A cosa sono serviti? Quali sono stati i risultati pratici di queste riunioni a Villa Pamphilj? Che fine hanno fatto le indicazioni e il programma della *task force* dell'ingegner Colao? La conferenza stampa finale si è conclusa con un invito al taglio dell'IVA, che dopo due giorni è già scomparso dai registri della politica. commentatori non di destra hanno detto che la cartella degli Stati generali è vuota e un altro famoso intellettuale di sinistra ha detto che sono stati gli Stati generali dell'aria fritta. Signor Ministro, io le chiedo: il piano di rilancio (*recovery

Presidente, come è noto e sarebbe bene che ci fosse un riconoscimento generale di un dato che appare oggettivo, l'Italia ha giocato un ruolo da protagonista nella definizione di una risposta europea ambiziosa alla crisi, che ha portato la Commissione europea a varare una proposta estremamente significativa che va esattamente nella direzione auspicata dall'Italia, come l'iniziativa *next generation* EU. EU. Intorno a questa opportunità il Governo ha deciso di varare un ampio ciclo di incontri, di consultazioni e di coinvolgimento di tutte le forze sociali e produttive del Paese, al quale sono state invitate a partecipare anche le forze di opposizione, che hanno scelto di non partecipare a incontri importanti, che si sono svolti peraltro in una sede istituzionale, esattamente come si sono svolti a Palazzo Chigi. Nonostante questo, il Governo ha reiterato l'invito a concorrere alla discussione sull'elaborazione di un ambizioso programma di rilancio dell'economia italiana. Come ho avuto modo di dire anche ieri in occasione dell'audizione alla Commissione bilancio della Camera, la presentazione e la discussione in Parlamento del Piano che il Governo presenterà e che già raccoglierà elementi emersi nel corso degli Stati generali, sarà auspicabilmente l'occasione di un confronto ampio con tutto il Parlamento sulle linee di fondo di una strategia di rilancio del Paese, che ha un'ambizione e una portata pluriennale e che intende non solo affrontare le conseguenze economiche del coronavirus, ma anche nodi e questioni strutturali di lungo periodo, che da troppo tempo hanno fatto dell'Italia un Paese che cresce meno degli altri Paesi europei, che ha un livello di occupazione troppo basso e diseguaglianze sociali e territoriali troppo alte, nonché un livello di investimenti inadeguato. Intorno a questa opportunità noi rilanciamo l'invito a tutte le forze responsabili a concorrere alla definizione di un piano ambizioso che l'Italia intende Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) a settembre, che definirà in modo dettagliato gli investimenti e le riforme che l'Italia intende varare nel quadro del programma europeo *next generation* EU, che invece porterà prima dell'estate a elaborare la cornice più ampia del quadro di riforme che il Governo intende realizzare nell'orizzonte di legislatura. La maggioranza ha indicato un chiaro orientamento anche nella predisposizione di quella cornice di piano di rilancio che è stata presentata a tutte le forze sociali e territoriali. Stiamo finalizzando il lavoro che troverà, come ho detto, nel PNR parte del suo documento concreto sottoposto al Parlamento. Rilanciamo l'invito a tutte le forze che hanno a cuore il futuro del Paese, e non le polemiche inutili che non interessano i cittadini, di concorrere con le loro idee alla definizione di un piano ambizioso all'altezza delle sfide che l'Italia ha davanti a sé. Signor Presidente, purtroppo la risposta non mi sorprende e mi delude perché ho la sensazione che anche il Ministro non sia così entusiasta di dover difendere gli Stati generali, ma questa è una mia maliziosa supposizione. Il fatto è che, ancora una volta, registriamo promesse vaghe e generiche, rimandi a settembre e all'estate, ma l'Italia, il nostro Paese ha drammaticamente bisogno di risposte urgenti, signor Ministro. Noi non ascoltiamo, non percepiamo una lista precisa di idee chiare e distinte, di scelte coraggiose da fare oggi, subito,

che noi non possiamo attendere oltre, né possiamo tollerare che le passerelle a Villa Pamphilj sostituiscano la politica, le scelte e il coraggio. Noi vorremmo sapere che cosa vuol fare questo Governo, quando intende farlo, con quante risorse, con quali risorse, se ci saranno denari che proverranno dall'Unione europea o saranno ancora una volta solo promesse e in quanto tempo intende assolvere a questi programmi urgenti. Di annunci ne abbiamo sentiti anche troppi. Noi, come posizione, come Gruppo Fratelli l'Italia, siamo ancora una volta disponibili al confronto nelle sedi istituzionali dove faremo come sempre il nostro dovere.

Signor Presidente, signor Ministro, quando si parla di condizioni materiali delle persone, di quella gigantesca questione sociale che rischia di abbattersi sul nostro Paese, una premessa d'obbligo: non c'è politica che possa garantire la dignità delle persone che non passi attraverso politiche che assicurino alle stesse lavoro e occupazione, perché il lavoro resta comunque l'elemento fondante dell'identità sociale delle persone e il lavoro si crea con politiche per lo sviluppo, politiche industriali, politiche per l'occupazione. Non vi è dubbio, Ministro, che siamo entrati in una fase della storia del mondo - lo dico con un certo pudore visto che sto parlando a uno storico

che le persone possono perdere quel lavoro nel giro di pochissimo tempo, che quel tratto di precarietà, di intermittenza e di fragilità di molte carriere lavorative rischia di diventare drammaticamente cronico e, a fronte della molteplicità di figure professionali che rispondono ad una molteplicità di configurazioni contrattuali, esiste oggi una molteplicità di misure e di strumenti di sostegno al reddito, di ammortizzatori che - ahimè - rischia, proprio a causa della frammentarietà, di mettere sul terreno un elemento di disparità e disuguaglianza e addirittura di aumentare i divari preesistenti. Se facessimo l'elenco delle categorie - che poi vuol dire delle persone - che rischiano di non essere comprese nelle maglie larghe degli ammortizzatori esistenti, nonostante i grandissimi sforzi che già questo Governo sta mettendo in campo a partire dai primi decreti per contrastare l'emergenza, pensare ai precari, agli esodati, agli stagionali, ai lavoratori delle cooperative sociali, a quel mondo che si è mobilitato in queste settimane dei lavoratori dell'arte, della musica, della cultura

del nostro Paese e, dall'altro, non ci curiamo di chi quella bellezza la valorizza quotidianamente col proprio lavoro. Voglio dire che penso sia arrivato il tempo di iniziare ad asciugare gli strumenti che esistono già e di immaginare - credo che questo debba essere lo sforzo del Governo una sorta di ammortizzatore universale. Non mi impicco alle etichette, ma siamo entrati in una fase nella quale questa deve essere la novità del tempo nuovo. Ci dobbiamo confrontare su questo tema immediatamente, con le misure

le competenze dirette del Ministero del lavoro ma che, per la sua portata, investe e interessa tutto il Governo e tutta la maggioranza. Correttamente si è ricordato come di fronte a una crisi senza precedenti come quella causata dal coronavirus, il Governo si è adoperato con strumenti straordinari per garantire, nella specificità e nella diversità degli strumenti, l'universalità di un principio, quello di sostenere tutti i lavoratori attraverso la cassa integrazione per tutte le tipologie di lavoratori dipendenti e strumenti nuovi come le indennità per i lavoratori autonomi parasubordinati e le altre tipologie. è anche istituito il reddito di emergenza, per supplire a situazioni particolari, non coperte da uno strumento pure significativo e di grande portata universale,

È del tutto evidente che questa esperienza, ma anche le trasformazioni più generali a cui il senatore interrogante faceva riferimento, pongono il tema non solo di affrontare la situazione di emergenza, per tornare semplicemente allo *status quo ante*,

Sarebbe opportuno, in questo quadro, chiarire meglio la distinzione tra strumenti di contrasto alla povertà e strumenti legati invece alla disoccupazione e alle politiche attive del mondo del lavoro.

che egli abbia posto un tema importante e invito pertanto le forze della maggioranza innanzitutto, ma tutto il Parlamento, a misurarsi sulla sfida a cui ha fatto riferimento, che vede il Governo impegnato a trarre lezioni da un tempo che cambia, per rilanciare, nelle forme nuove, i principi di universalità del *welfare* e di sostegno al lavoro. Signor Ministro, la sua risposta ci indica che il Governo è attento alla questione che abbiamo posto e sta lavorando esattamente nella direzione che auspichiamo.

che quel lavoro si può distruggere da un momento all'altro e che ci vuole del tempo a ricostruirlo e quindi penso che alcuni tabù debbano essere rimossi, come penso che i provvedimenti di cui ci stiamo occupando e di cui ci occuperemo debbano essere informati da un principio, il massimo della condizionalità delle misure destinate alle imprese - alle imprese bisogna infatti dare molti soldi, ma occorre vincolarli alla difesa del perimetro occupazionale e agli investimenti: questa è la condizione che dobbiamo porre - e il massimo dell'universalità delle misure destinate alle persone, perché le condizionalità non siano un

che a partire da questa maggioranza e da questa esperienza di Governo costruissimo uno Stato che lanciasse il suo *«whatever it takes*» alle persone, che vuol dire impedire che le persone caschino nel vuoto, quando quel vuoto si dovesse determinare. Sarebbe un fatto di civiltà, un fatto di dignità e, sicuramente, un elemento di

Ministro, sappiamo che la pandemia non è stata soltanto una crisi, ma una vera e propria rottura di civiltà. Abbiamo avuto un problema, riguardante il nostro sistema delle imprese, che "cuba" questi numeri: milioni e 300.000 piccole e medie imprese, che davano luogo a 15 milioni di persone occupate, sono a rischio un milione di piccole e medie imprese, con tre milioni di occasioni di lavoro. Abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo risorse importanti sia come sistema Paese, sia nel dialogo competitivo con l'Europa: 80 miliardi già in esercizio e quelle che sono ulteriormente assumibili. Abbiamo priorità che si aggiungono a quelle precedenti alla crisi e alla rottura di civiltà. Dobbiamo fare in modo che sia facile la vita delle imprese; dobbiamo mettere in campo un piano delle infrastrutture che non sia da convegnistica, ma che sia capace di migliorare la vita delle persone, delle imprese e dei territori; dobbiamo fare in modo di liberare il reddito da lavoro per quanto riguarda la pressione fiscale; dobbiamo ricostituire e ricomporre il bilancio pubblico del nostro sistema Paese. C'è bisogno di mettere in campo una riforma organica del sistema fiscale e tributario, lo ha detto anche ieri il vertice della Corte dei conti, sia nella parte della procura generale, sia nella parte del Presidente delle sezioni riunite, che hanno conclamato che c'è urgenza di una riforma dal punto di vista fiscale e tributario. Abbiamo due numeri che ci guidano ancora di più, sapendo che il lavoro è in corso e dev'essere rafforzato, supportando la sua iniziativa: 110 miliardi di euro di evasione fiscale 210 miliardi di economia sommersa. Lo ha detto prima: abbiamo un credito scritto nei documenti contabili, per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate-Riscossione, pari a 950 miliardi di euro. Ha detto che vuole farsi carico, come ha richiesto anche il direttore generale dell'Agenzia delle entrate, di ridurre questo credito a un ottavo, che nei fatti equivale realmente a 110 miliardi di euro. euro. Dobbiamo lavorare per far sì che le 800 leggi e norme che riguardano il nostro ordinamento tributario conoscano una semplificazione, una *reductio ad unum*, in modo che l'ordinamento tributario sia una funzione per l'adempimento dell'articolo 53 della nostra Carta costituzionale. Dobbiamo fare in modo anche che i 47 milioni di euro scritti nella legge di bilancio nella legge di bilancio in esercizio, per dotare di ulteriori risorse umane e tecnologiche le nostre agenzie fiscali, vengano subito messi in produzione, perché abbiamo bisogno di potenziare la macchina, proprio per mettere mano ai problemi che sono stati segnalati, e la legge di bilancio a tale proposito rappresenta un punto fermo di riferimento. C'è bisogno, signor Ministro, di conoscere le iniziative che assumerà per far sì che con quell'articolo 71 del decreto cura Italia, in cui per la prima volta si parla di premialità fiscale, chi adempie agli obblighi fiscali in questa stagione di rottura, di pandemia e di crisi della civiltà vada riconosciuto e premiato, così come va aiutato chi non ce la fa. però adempie e dà luogo all'obbligo dell'articolo 53 dev'essere riconosciuto per la sua virtù, perché anche su questo si fonda e vive un ordinamento nazionale. Dobbiamo creare lo spazio fiscale unico europeo, anche per agire in sede europea rispetto, ad esempio, alla *web tax.*

di facilità e di un patto di fiducia tra cittadino contribuente, impresa e ordinamento. Sappiamo che si può fare e conosciamo la volontà e la motivazione: mettiamoci insieme e ci riveli i tempi per questa straordinaria operazione.

la riforma fiscale e tributaria e anche il ruolo dell'amministrazione finanziaria, per rendere concreto quel patto di semplicità cui ha fatto riferimento e un modello di cooperazione con il contribuente basato sulla trasparenza, sulla semplificazione, sulla razionalizzazione degli adempimenti e sulla qualità dei servizi. Da questo punto di vista, vorrei anche sottolineare l'impegno che l'Agenzia delle entrate sta profondendo in tale direzione, anche temporaneamente - e questo è un elemento della premialità a cui faceva riferimento - trasformandosi in agenzia delle uscite, con un livello di efficienza degno di nota, visto che ieri sono partiti i bonifici dei contributi a fondo perduto, in anticipo sulla tabella di marcia, sulla base di una procedura semplice ed efficace, che si sta rivelando molto positiva. Quindi un'amministrazione finanziaria che investe sull'innovazione e sulla digitalizzazione può rafforzare il suo rapporto positivo con i cittadini e anche svolgere compiti nuovi in una fase di emergenza che poi magari, dal punto di vista della tecnologia

e alla concreta esigenza, che il Governo intende affrontare, dell'eliminazione dal magazzino dell'Agenzia di queste pratiche creditorie solo nominali, per rafforzare invece la capacità di riscossione, dove effettivamente ci sono margini per recuperare imponibile per le casse dello Stato. Più in generale, l'obiettivo è quello di creare un *business climate* favorevole per riconoscere maggiore competitività alle imprese italiane e favorire l'attrattività di investimenti delle imprese nel territorio nazionale. quindi di un ampio *set* di misure che vanno affrontate nel quadro di una riforma più generale di un fisco più equo, rispetto alla quale - e qui integro la risposta alla senatrice Conzatti - c'è il tema della rivisitazione delle *tax expenditure*, una razionalizzazione delle quali, dal punto di vista strutturale, può liberare risorse molto importanti per una riduzione delle aliquote. Infine, ha fatto riferimento a una misura molto significativa che il Governo ha varato

che è impegnato nel rafforzamento della misura. Prima di passare a una sua attuazione, ci è sembrato corretto, vista la richiesta del Parlamento di rafforzare ulteriormente la misura, attendere l'esito del confronto parlamentare, per poi rendere operativa una misura che auspichiamo possa dare un contributo significativo, non solo al rilancio dell'economia, ma anche alla sua qualificazione dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dell'efficienza energetica e della capacità di riduzione del rischio sismico.

Ha indicato i pilastri fondamentali di una riforma fiscale e credo che sia molto importante anche riconoscere al nuovo ruolo che ha assunto l'Agenzia delle entrate un particolare rilievo, perché rappresenta, per efficienza e semplicità, la condizione fondamentale per stabilire un nuovo rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini proprio nella semplificazione, nella velocità e nell'efficientamento del sistema del nostro Paese. Siamo assolutamente consapevoli dell'esigenza di una nuova riforma fiscale come pilastro fondamentale per accompagnare una nuova idea dello sviluppo economico del nostro Paese. Essa dev'essere ispirata a principi di equità e progressività; deve ristabilire un rapporto più positivo e più proficuo nelle relazioni tra lo Stato e i cittadini; deve ispirarsi a processi di razionalizzazione ed efficienza. L'abbiamo già dimostrato: in poco tempo, abbiamo consegnato alle nostre spalle, quasi come relitti della storia, sia i condoni fiscali sia una visione sovranista degli Stati che contrastano la dimensione europea. Abbiamo di fronte a noi una grande opportunità, un nuovo volto dell'Europa, non solo in termini quantitativi per le risorse a disposizione. Abbiamo cioè le condizioni per uscire da una narrazione al passato, anche grazie alle misure introdotte per superare l'emergenza, e costruire una dimensione economica per il futuro del nostro Paese. In tutto questo c'è anche una grande opportunità,

Ritengo pertanto che tutto questo sia una straordinaria opportunità per far sì che la nuova riforma fiscale possa rappresentare un pilastro fondamentale per garantire velocità, efficienza e anche premialità alla fedeltà fiscale, che rappresenta inevitabilmente una condizione per favorire e agevolare nuovi investimenti delle imprese, orientandole verso il futuro, la *green economy* e e l'economia digitale, fondamentale per costruire il nuovo sviluppo economico. Credo che ciò abbia bisogno di una riforma fiscale adeguata, che velocizzi e produca nuovi investimenti per il futuro del nostro Paese

L'attuale quadro economico rende tale disparità ancora più preoccupante: è necessario un vero piano di rilancio affinché tutto il Paese riparta e l'infrastrutturazione del Meridione è condizione essenziale perché ciò avvenga. Non mi stancherò mai di ripetere che la nostra economia non potrà mai rialzarsi senza il Sud, signor Ministro, e senza la valorizzazione delle sue enormi potenzialità. Se il Governo non avvierà al Sud una crescita capace di autosostenersi, il Paese non uscirà dal guado. In tale contesto, il ponte sullo Stretto di Messina, oggi come non mai, rappresenta un'opera strategica, che garantirebbe non solo la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d'Italia, ma anche quella tra il nostro Paese e il resto d'Europa, comportando grandi vantaggi in termini di sviluppo economico e sociale, oltre che di immagine. Esponenti della maggioranza e rappresentanti del Governo, come il ministro De Micheli, appena una settimana fa in quest'Aula hanno mostrato interesse nella realizzazione dell'opera. Finalmente si sta iniziando a comprendere che infrastrutture di tale portata consentirebbero non solo di creare nuovi posti di lavoro e di riattivare il tessuto economico, ma anche di attrarre investimenti, trasformando la crisi in un'opportunità di sviluppo. Il ponte rappresenta anche una potente attrattiva turistica: pensiamo alla quantità di turisti richiamati dai ponti più spettacolari e suggestivi del mondo. Iconico è il ponte sullo stretto di Akashi, in Giappone: 22 milioni di turisti l'anno pagano un biglietto di 27 euro per ammirare il panorama mozzafiato che si gode dalle sue torri. Le assicuro, signor Ministro, che la vista dall'alto dello stretto di Messina sarebbe altrettanto spettacolare. Per tutti questi motivi, Forza Italia da sempre sostiene l'importanza del ponte. L'ultimo Governo Berlusconi aveva avviato la realizzazione del progetto, bloccato poi dal Governo Monti, e tale decisione sta costando svariati milioni agli italiani, un dispendio inutile di danari pubblici, che avremmo potuto investire in modo proficuo e che invece stiamo gettando al vento. L'Unione europea, come ben sa, ha più volte sollecitato l'Italia

qui un articolo del «Corriere della sera» del 1985, che titolava sul via libera al ponte sullo Stretto e annunciava il completamento dell'opera nel 1995; la storia poi la conosciamo. Entrando nel merito, uno dei problemi fondamentali è derivato dal fatto che un'opera di questa portata e anche di queste potenzialità per lo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno esige naturalmente una rigorosa valutazione di sostenibilità economico-finanziaria in relazione al costo aggiornato del progetto definitivo. Il costo originario del progetto a cui lei fa riferimento ammontava a quasi 6 miliardi di euro, a cui se ne aggiungevano oltre 4 di opere compensative richieste dai territori. Il costo complessivo dell'opera nel 2012 non ne consentiva quindi la sostenibilità finanziaria nella modalità allora contrattualmente prevista. Per tali motivazioni, il progetto non ebbe corso e il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 dispose la liquidazione della società,

Come ha ricordato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sta ora valutando la percorribilità della realizzazione del ponte nell'ambito di una stringente *project review* che riduca drasticamente il costo del progetto definitivo, anche al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria. Si terrà conto degli esiti di una puntuale analisi costi-benefici e del dibattito pubblico cui verrà sottoposto il progetto, valutando altresì le ricadute in termini occupazionali, ambientali e trasportistici alla luce degli investimenti infrastrutturali già programmati nel territorio siciliano e di tutti i profili giuridici connessi al contenzioso in corso con il soggetto attuatore e il *general contractor.* Tali valutazioni sono ovviamente propedeutiche alla ricognizione delle possibili fonti di finanziamento, rispetto alle quali, naturalmente, le nuove risorse europee costituiscono una fonte su cui è opportuno fare una valutazione.

dei Paesi frugali solo presentando alla Commissione europea progetti credibili e dettagliati per ammodernare il Paese, nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, come sa bene. Non perdiamo tempo: facciamolo subito ed evitiamo gli errori del passato. Ai detrattori dell'opera, che a giustificazione dei loro no portano la necessità di dotare prima il Sud di una rete ferroviaria adeguata e di strade, autostrade e porti moderni, dico che si nascondono dietro un alibi che ha paralizzato per anni ogni iniziativa a favore dei meridionali. La costruzione del ponte attiverebbe finalmente un circolo virtuoso di investimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno, che andrebbe a connotarsi come polo logistico dell'Italia e dell'Europa. Sebbene l'Unione europea continui a chiederci politiche economiche basate su investimenti strategici, negli ultimi anni il Meridione è stato totalmente abbandonato. Dei circa 63 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, solo solo una minima parte è stata utilizzata (parliamo del 3-4 per cento). Questo Governo ha destinato fin troppe risorse alla ricerca del consenso elettorale, dimostrando di non saper investire nel futuro del Paese. Non si può continuare a governare distribuendo prebende e *bonus*, pensando solo a salvaguardare le proprie poltrone e ignorando il costo che le generazioni future pagheranno per tali politiche. Il tempo è scaduto. Il *recovery fund* potrà essere un'occasione per invertire la rotta, ma non dobbiamo lasciare nulla al caso e soprattutto dobbiamo partire dall'assunto per cui il Sud non può più essere trattato come una zavorra, ma rappresenta il motore da accendere per far ripartire l'Italia intera.

Signor Ministro, nella nostra interrogazione ci siamo permessi indegnamente di storicizzare, per lei che è uno storico, le vicende degli ultimi centododici partendo da quando, il 5 marzo, presentaste una relazione che chiedeva - con nostro sbigottimento - uno scostamento di appena 6,35 miliardi e arrivando agli attuali dati, che ci raccontano come, a fronte di 62,9 miliardi di acquisti di titoli italiani da parte della BCE, le emissioni nette del Tesoro siano state di appena 57,9 miliardi. Non so se, leggendo queste premesse, si è reso conto del disastro che avete combinato. Le regole vogliono che l'interrogazione sia contenuta in una pagina, ma la nostra si sarebbe potuta riassumere in una parola: perché? Perché non ci avete ascoltato, quando vi abbiamo detto che lo scostamento da votare doveva essere all'altezza della tragicità della situazione e che avremmo dovuto fare come la Francia, che in occasione dell'ultima, meno grave, crisi globale aveva risolutamente scelto di espandere il *deficit* fino al 7 per (138 miliardi di euro), non solo per contenere i danni immediati, ma soprattutto per gestire meglio il rapporto con i fratelli europei, che possono scusare un *deficit* alto in circostanze eccezionali, purché poi lo si diminuisca? Vi abbiamo spiegato anche che il finanziamento di questo *deficit* non era un problema, perché era chiaro che la BCE non aveva alternative: o espandere il suo ombrello o far saltare le banche francesi e tedesche e quindi l'euro. Bisognava quindi procedere emettendo titoli di Stato, che avrebbero incontrato il favore dei risparmiatori italiani, e bisognava farlo subito; lo avete fatto dopo, il 16 maggio. Perché? Perché voi, che siete così ben visti e ben introdotti nei salotti europei, dove i TG vi ritraggono scodinzolanti, ci avete messo venti giorni ad approfittare delle nuove norme sugli aiuti di Stato (la Francia solo quattro) e quaranta giorni ad approfittare della sospensione del Patto di stabilità con un nuovo scostamento (la Germania solo tre)? Perché? Queste reazioni ovvie vi hanno colto di sorpresa? I vostri amici europei non ve ne avevano parlato? Oppure sapevate, ma avete voluto cogliere l'occasione per eliminare i vostri nemici di classe? Un secolo dopo, eliminare i *kulaki* è ancora una priorità, a quanto pare, che oggi sono i professionisti lasciati senza indennità, i piccoli e medi imprenditori senza credito, ma anche gli operai senza cassa integrazione. O forse volevate solo consolidare il vostro potere, costringendo il Paese a entrare in patti leonini, come il MES, con istituzioni governate da nostri avversari economici che sono vostri alleati politici? Perché, ma anche quanto? Quanto sarà il prossimo scostamento? Quanto ci costeranno i vostri ritardi? La risposta, signor Ministro, ci interessa non solo dal punto di vista politico, ma anche umano e storico. La più grande catastrofe della storia economica italiana ha un nome,

L'interrogazione dimostra con ogni evidenza una non piena conoscenza - o forse una scarsa conoscenza - dei meccanismi e delle tecniche di emissione del debito pubblico. *(Applausi)*. Vorrei concentrarmi su questi aspetti, non non sul resto, che è abbastanza evidente ed oggettivo: l'Italia ha realizzato lo sforzo di politica di bilancio maggiore in Europa, secondo solo a quello della Germania, per far fronte al coronavirus.

agli acquisti della Banca centrale europea), cerco di andare con ordine. È noto ed evidente che lo sforzo è stato senza precedenti, ampliando la portata dei meccanismi di collocamento esistenti, creandone di ulteriori e mettendo in campo anche nuovi strumenti. In pochissimi giorni, il Dipartimento del tesoro ha saputo porre in campo una strategia che ha consentito all'emittente di aumentare da subito e in modo molto significativo la provvista finanziaria con modalità compatibili con le condizioni di mercato e con la gestione dei rischi di tasso e di rifinanziamento. Come dicevo, l'interrogazione parte da presupposti non corretti. luogo, non appare corretto prendere come riferimento l'ammontare di acquisto di titoli italiani da parte della BCE, in quanto si tratta di riferimento indiretto, relativo al mercato secondario, non potendo tale istituzione fare acquisti direttamente su quello primario; un confronto diretto appare fuorviante e, in ogni caso, non possono che essere cifre parziali rispetto a quelle programmate dai Paesi come collocamenti di titoli.

È forse opportuno ricordare che, nella prima metà del mese di marzo, per effetto dell'esplodere delle conseguenze della pandemia, prima in Italia e poi nel resto d'Europa, le condizioni di mercato dei titoli di Stato erano divenute più difficili. Un aumento importante delle emissioni già da inizio marzo, oltre al fatto di non avere alcun fondamento in base alle previsioni di raccolta di allora, non avrebbe fatto altro che aggravare ulteriormente condizioni di mercato già particolarmente difficili. L'altro presupposto non corretto, anche volendo fare un confronto diretto tra emissioni e programma di acquisti della BCE, è che questo venga fatto in termini di emissioni nette, dal momento che sono quelle lorde a rappresentare le reali esigenze di copertura del fabbisogno statale, comprensive, cioè, delle scadenze di titoli, che evidentemente l'interrogante si è dimenticato di conteggiare. Le emissioni nette risentono del profilo dei rimborsi e ciò rende il paragone poco significativo. Venendo alle cifre, nel periodo da marzo a maggio 2020, si sono avute emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine pari a 117,26 miliardi di euro, esclusi i BOT, pari a 56,7 miliardi in termini di valore nominale. Nello stesso periodo del 2019, le emissioni lorde a medio-lungo termine furono pari a 65 miliardi circa, cui vanno aggiunti 39,1 miliardi di BOT. Le maggiori emissioni a medio-lungo termine in questo trimestre sono state quindi di 52,26 miliardi e i BOT sono aumentati di 17,6 miliardi rispetto all'anno precedente. Facendo un confronto da inizio anno e fino al 15 giugno 2020, si sono avuti 92,7 miliardi di maggiori emissioni rispetto al 2019, con un incremento del segmento a medio-lungo termine di 76,9 miliardi e di 15,8 miliardi con riferimento ai BOT. Si fa altresì presente che nella nota di aggiornamento al DEF dello scorso anno si prevedeva un fabbisogno di circa 45 miliardi di euro. Pertanto, in termini di emissioni lorde, era previsto un totale di circa 247 miliardi di euro, pari ai citati 45 miliardi di fabbisogno, più 202 miliardi di scadenze a medio-lungo termine. A maggio sono stati emessi ben 171 miliardi di euro di titoli a medio-lungo termine, che rappresentano circa il 70 per cento di quanto era stato previsto di emettere per il 2020 a fine 2019. A queste cifre, va aggiunto l'ammontare di titoli a breve termine BOT, che sono stati emessi a oggi per un ammontare superiore a quelli in scadenza di oltre 20 miliardi e che hanno costituito ulteriore fonte di finanziamento netto, a fronte di una stima a fine 2019 di emissioni nette di BOT nulle. Risulta pertanto chiaro lo sforzo senza precedenti condotto per far fronte alle aumentate esigenze di raccolta emerse nel corso degli ultimi mesi e risulta altrettanto evidente lo scarso fondamento empirico

Signor Ministro, secondo la liturgia parlamentare ora dovrei dirle di non essere soddisfatto della sua replica, ma mentirei: sono soddisfattissimo. Il *question time* è come la lanterna di Diogene e non cercavamo la spiegazione di una dinamica economica che abbiamo capito prima e meglio di lei, tant'è che alla fine i fatti ci hanno dato ragione. Sta facendo tardi e male ciò che avevamo chiesto di fare presto e bene, cioè 100 miliardi di scostamento per interventi immediati, finanziati con titoli rivolti prevalentemente ai risparmiatori italiani. (*Applausi*). Quanto sia lo scostamento prossimo - cioè, il costo dei suoi ritardi - non ce lo ha detto, ma va bene così, perché cercavamo l'uomo e l'abbiamo trovato: una mistura di rifiuto della realtà, supponenza verso il Parlamento e tanto amore per il burocratese. Non è corretto dire che lo sforzo italiano è il più ampio o, come ama dire, il più ambizioso,

nato per far eleggere al Parlamento un Presidente della Repubblica a immagine e somiglianza della sinistra, non solo non ha in Parlamento una maggioranza solida per condurre a termine questo scippo istituzionale, ma nella Camera alta le comunico che non ha nemmeno la maggioranza assoluta per farsi votare il prossimo necessario scostamento, su cui lei non ci ha informati. (*Applausi*). Mi permetta allora di darle un consiglio costruttivo: deponga la sua arroganza, si adoperi per una vera condivisione e ascolti chi ne sa più di lei, come i tanti parlamentari della Lega che in questi tre mesi, con dedizione e patriottismo, hanno cercato di farle intendere ragione. Deleghe in bianco non ne daremo più: buon lavoro.

*(M5S)*. Signor Presidente, nelle classifiche internazionali l'Italia è ai primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà d'informazione: due facce della stessa medaglia.

infetta». Questa malapianta, difficile da estirpare (analogamente alle raccomandazioni), coinvolge purtroppo tutte le categorie sociali, economiche e istituzionali. In molte delle 60.000 intercettazioni della maxi-inchiesta maxi-inchiesta che ha travolto l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati Palamara per le presunte nomine pilotate di togati, oltre a un mercimonio della funzione giudiziaria, appaltata al sistema delle correnti, con forti dubbi su alcune sentenze non sempre equilibrate ed emesse secondo i canoni della giustizia uguale per tutti, emerge la rete di influenze e relazioni funzionali al sistema di raccomandazioni attivato per ottenere incarichi, che ha inferto profonde ferite alla magistratura.

medicina a Tor Vergata. Ebbene, si incontra con il rettore Novelli e arriva a vincere all'università di Tirana, previo appuntamento, dove si sarebbe presentato in compagnia della madre di Mancinetti *junior*, Anna Maria Soldi, sostituto presso la Corte di cassazione. Magistrati solerti, forse politicizzati, che, in barba all'articolo 68 della Costituzione, secondo il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, aprono indagini a tamburo battente su senatori, dopo la denuncia di un ex direttore generale, con l'utilizzo del nucleo della Guardia di finanza e dell'autorità a suo uso e consumo, rei di aver osato presentare atti di sindacato ispettivo sull'Agcom, dimenticando per circa due anni di istruire il procedimento dopo l'interrogatorio iniziale e certi dell'impunità della corrente. Se nella separazione equilibrata tra poteri dello Stato si fa prevalere la funzione giudiziaria, si ripete l'errore esiziale della politica, che ha delegato poteri ad oligarchi, facendo prevalere la finanza sull'economia reale; quel club esclusivo di persone non elette democraticamente che decide i destini del mondo dopo aver manipolato i mercati. Chiudo, signor Presidente, ringraziandola: le democrazie funzionano con pesi e contrappesi, i quali, se vengono meno, possono aprire varchi all'autoritarismo e impedire, con la famigerata circolare bavaglio, di chiedere conto, con atti di sindacato ispettivo, delle malefatte dei magistrati. Ci sono tante interrogazioni bloccate: significa mortificare la funzione e le prerogative dei senatori e infliggere un colpo alla dialettica democratica. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, in un articolo *on line* apparso sul sito www.key4biz.it dello scorso 16 giugno, si apprende che Zoom, *software* usato per organizzare videoconferenze, ne avrebbe censurate due organizzate dagli Stati Uniti (non dalla Cina) per la commemorazione dell'anniversario del massacro di piazza Tienanmen. Sappiamo che anche il Senato usa Zoom ed è utilizzato, in particolare, per le audizioni informali che si svolgono in Commissione. Questa piattaforma per videoconferenze di tipo commerciale, insieme ad altre, anch'esse commerciali, utilizzate dalla scuola per la didattica a distanza e dalla pubblica amministrazione per lo *smart working*, presenta diverse criticità per la tutela dei dati personali, per la robustezza dell'infrastruttura tecnologica e, come anzidetto, ci sono problemi anche di carattere politico. Infatti la funzionalità di censura automatica consente di dedurre che non c'è riservatezza sulle comunicazioni e che le videoconversazioni, come ammesso nelle *privacy policy*, possono essere utilizzate a scopo di profilazione. Le amministrazioni dello Stato devono prendere provvedimenti. Il Governo tedesco ha infatti proibito l'utilizzo di Zoom. Tuttavia queste problematiche non devono farci retrocedere nei passi compiuti in questi mesi verso la digitalizzazione del Paese, invece renderci sempre più consapevoli riguardo i retroscena che ci sono nell'utilizzo delle tecnologie. Le tecnologie digitali raccolgono dati e i dati sono la nuova materia prima per le applicazioni del futuro. Dobbiamo decidere se vogliamo continuare a regalare ai *competitor* queste materie prime o vogliamo iniziare a sfruttarle internamente. Le alternative alle piattaforme commerciali dei colossi extraeuropei esistono. Esistono le piattaforme *open source*. I colleghi spagnoli e francesi hanno già implementato la videoconferenza di Stato sia per la funzionalità degli uffici pubblici sia per la didattica a distanza. Occorre che lo facciamo anche noi. Nelle applicazioni della pubblica amministrazione che implicano il trattamento di dati personali, in particolare nelle applicazioni per la scuola, si dovrebbe vietare per legge l'uso di prodotti dei quali non sia conosciuto il codice sorgente. In Italia, come alternativa ai colossi commerciali, è partita l'iniziativa volontaristica di «iorestoacasa.work», basata sull'utilizzo di codici *open source* e attorno alla quale si sono raccolte le migliori professionalità informatiche uscite dalle nostre università. Per realizzare il progetto sono state

perché le istituzioni italiane hanno finora preferito sistemi privati e proprietari fuori dal loro controllo, invece di utilizzare soluzioni aperte, pubbliche e controllate da loro? Ne aggiungo un'altra mia: perché le decisioni su acquisti e soluzioni riguardanti la digitalizzazione dei servizi pubblici non sono nelle disponibilità dei nostri migliori esperti, ma sembra dei peggiori? Non lo dico solo io, anche il professor Angelo Raffaele Meo nella sua recente lettera alla ministra Azzolina, sottoscritta dalle associazioni del *software* denuncia le scelte scellerate degli ultimi decenni. Il nostro Paese è praticamente uscito dal comparto industriale delle tecnologie dell'informazione. Nella lettera si chiede una legge che proibisca l'uso di *software* proprietario nelle applicazioni della

negli ultimi anni. Abbiamo milioni di progettisti e programmatori che possono essere un'importante opportunità per l'economia del nostro Paese ed è opportuno destinare gli investimenti che verranno a breve realizzati nel digitale esclusivamente a tecnologie in *software* libero. Le proposte e le alternative quindi ci sono e mi auguro che anche il Senato, la scuola e tutta la pubblica amministrazione possano adoperarle nel più breve tempo possibile. Siamo chiamati alla transizione digitale da percorrere in tempi ridotti; facciamolo decisamente puntando sulle nostre risorse. Sovranità digitale significa mettere a sistema i nostri cervelli, le nostre infrastrutture

Per il resto, invece, come molte istituzioni pubbliche, anche il Senato utilizza le piattaforme comuni di mercato. I suoi rilievi sono articolati. Sarà cura della Presidenza segnalarli